il provvedimento, il cui iter in Commissione si è concluso il 1º febbraio 2017, è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea 31 maggio 2017 per un nuovo esame, in quanto la Commissione Bilancio non si è potuta pronunciare in senso favorevole sul testo a seguito di alcuni rilievi critici

del 6 giugno è stato evidenziato che l'istruttoria sul testo non si riteneva ancora completata e soddisfacente in quanto la Ragioneria generale dello Stato richiedeva una ulteriore relazione tecnica al Ministero del lavoro, ritenendo la precedente incompleta e non scevra da criticità; del 20 giugno sono state segnalate forti criticità nel testo: *a)* le ulteriori correzioni del Relatore, approvate in Commissione, finalizzate a superare i rilievi della Commissione Bilancio e della Ragioneria generale dello Stato, volte a garantire l'effettiva invarianza finanziaria del provvedimento, rendono il testo, privo di adeguate risorse finanziarie, una mera dichiarazione di intenti; il provvedimento disattende le aspettative delle persone sorde. Infatti, il disegno di legge, già contrastato dalle persone sorde sostenitrici del metodo oralista, le Amministrazioni interessate non saranno in grado di provvedere in maniera efficace all'attuazione delle disposizioni introdotte nei limiti delle risorse umane, strumentali

segno che le sei legislature precedenti arrivarono alla conclusione che riconoscere la LIS non è il principale diritto delle persone con disabilità uditiva. Non dimentichiamo che il titolo iniziale di questo disegno di legge prevedeva il riconoscimento della LIS come minoranza linguistica: un abominio. L'incostituzionalità era del tutto evidente:

cioè una comunità fondata su origini, tradizioni, siti geografici , mentre si voleva riconoscere la LIS come minoranza linguistica, come se i disabili uditivi fossero una comunità isolata, contro la nostra Costituzione e contro tutti i diritti fondamentali riconosciuti alla disabilità di cui l'inclusione è il cardine (vedi l'atto votato il 14 settembre dal Parlamento europeo). È utile ribadire che l'acquisizione della parola è la premessa fondamentale per favorire processi di inclusione finalizzati alla piena cittadinanza e a questo s'impone prioritariamente un impegno congiunto delle istituzioni per concretizzare questo diritto attraverso la programmazione dei centri regionali per la diagnosi precoce attualmente attivi in poche Regioni italiane nonostante i LEA. Ritenere di risolvere l'*handicap* con un approccio limitato condanna la persona sorda a forme subdole di emarginazione che non giovano al successo scolastico e tantomeno alla piena cittadinanza.

Ora ci troviamo a discutere ed approvare probabilmente una scatola vuota, un'altra bandiera da sventolare. Mi è stato detto dal relatore, che ringrazio per il video commovente che ha inviato a tutti noi per dirci "ti voglio bene" nella lingua dei segni, visto che non ci sono oneri per lo Stato perché non approvare una legge che ormai serve solo a sottolineare i diritti delle persone disabili uditive? Io mi chiedo da quando il Parlamento fa leggi che servono a ribadire un'altra legge che già viene ampiamente applicata, la prima in Europa e forse nel mondo, la n. 104 del 1992 che garantisce - non promuove come viene detto in questo testo - una una uguaglianza formale e sostanziale alle persone disabili uditive che utilizzano la LIS o altri mezzi di comunicazione, e cioè:

cui le tutele previste da questa legge non venissero garantite, è possibile richiedere immediatamente la tutela giurisdizionale ai sensi della legge n. 67 del 2006. Quindi, quando l'ENS, che ha un buco di bilancio di almeno 12 milioni di euro, anche con accuse di appropriazione indebita dei Presidenti precedenti, continua a mandare lettere sottolineando come un cittadino sordo che deve fare denuncia alla polizia deve poter disporre di un interprete messo a disposizione dalle istituzioni o in ospedale o a scuola o vuol far assumere in tutto il servizio pubblico, ovunque, gli interpreti che promuove e forma o li vuol fare assumere e di conseguenza togliere il sussidio di indennità a 43.000 persone che lo ricevono in Italia, secondo i dati dell'INPS. infatti che ci sia sempre una questione di soldi dietro questo disegno di legge che dà disponibilità agli enti locali di provvedere, visto che la Ragioneria di Stato soldi non ne dà, o almeno ne sono stati dati garbatamente,

È da anni che il Nomentano aspetta di essere regolamentato dal MIUIR e si trova in un limbo, ma nel 2000 ha chiuso l'attività scolastica perché l'ha trasferita all'istituto Margarotto. Certamente c'è uno sportello che dà assistenza alle persone disabili ed per questo ci sono le ASL ed i centri preposti e soprattutto molti disabili uditivi non vogliono avere a che fare con questi.

e dare magari il milione di euro alle Regioni per implementare lo *screening* neonatale nei LEA? Non era meglio utilizzarli per la prevenzione e comunicazione di malattie infettive in gravidanza (quelle del sistema TORCH) che sviluppano sordocecità

quale lingua dei segni? Certo, c'è la lingua dei segni italiana, ma sappiamo che in Italia quasi ogni città ha delle varianti e che ci sono circa

come mai ancora oggi la logopedia, necessaria per processi abilitativi o riabilitativi per lo sviluppo del linguaggio, sia accessibile solo ai più fortunati o ai più abbienti, perché garantita a macchia di leopardo sul territorio nazionale o come prestazione privata a pagamento? Non è meglio indirizzarci verso le tecnologie e sviluppare la ricerca scientifica per contrastare la sordità? Ciò nonostante, ancora oggi nel Parlamento italiano assistiamo ad una controversa e annosa discussione sulla lingua dei segni, che risulta, oggi più che mai, una scelta ideologica fuori dal tempo, fuorviante fuorviante rispetto alle vere difficoltà che quotidianamente incontrano le persone con sordità o pluridisabilità. Serve invece una coerente azione di Governo improntata a diritti umani e costituzionali che, lungi da nuove leggi dal contenuto anacronistico, predisponga programmi triennali volti ad assicurare il diritto alla parola, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e alla comunicazione autonoma e uguale per tutti. *(Applausi

delle sensazioni più belle che accompagnano circa un milione di persone in questo Paese e che aspettano da un po' di tempo una risoluzione e un provvedimento di questo tipo, che le metta in condizione di poter ben

giovanissimi imparano a comunicare, e a chi magari non ne ha avuto la possibilità negli anni ed è diventato ormai adulto, di poter interagire con un apprendimento serio.

circa un milione di persone interessate (960.000, per la precisione); ma dovremmo probabilmente collegare ad esse anche tutte le famiglie. Vent'anni di ritardo - lo ha detto il relatore qualche mese fa

È vero, non c'è una legge che si occupi dei non udenti, ma è altrettanto vero che nel 1992, come ha ricordato il senatore Malan, c'era già un qualcosa che si occupava della disabilità in generale; forse in quel momento eravamo un po' troppo avanti. La storia dell'educazione dei sordi, anzi dei sordomuti, è sempre stata attraversata da forti polemiche su molte questioni, tra cui in particolare quella sull'uso dei metodi. Sono stati inventati e attualmente sono proposti i più disparati metodi, ognuno dei quali veniva e viene considerato spesso risolutivo della problematica. problematica. La contrapposizione più forte per le diverse implicazioni educative, linguistiche, culturali e sociali è stata quella tra il metodo orale e quello che, per semplicità, chiameremo gestuale. l'apertura del relatore qualche mese fa quando, all'inizio del suo intervento, ha parlato con

la composizione delle frasi sono assolutamente incredibili sotto l'aspetto grammaticale, sintattico, morfologico e lessicale. La LIS è una delle tante lingue dei segni diffusa in tutto il mondo, su cui esiste ormai una considerevole letteratura, che ci dice come quei segni, quei movimenti sono parole, affermazioni; insomma, sono Un concetto comune tra udenti è che la comunicazione tra sordi - probabilmente la battuta mi verrebbe facile, soprattutto nelle Aule parlamentari - sia diversa da quella che avviene considerandola una comunicazione povera, inferiore, che non ha la possibilità di spiegare magari concetti nobili piuttosto che complessi o di alta cultura.

In questo modo si aiutano i bambini a rapportarsi con i coetanei sordi, ad approcciarsi a uno strumento comunicativo in più. La LIS è una lingua a tutti gli effetti: si fanno letture, si insegnano i canti, le preghiere, e i bimbi riescono a costruire vere e proprie frasi compiute. La lingua dei segni non è una forma abbreviata di italiano, non è assolutamente una mimica né un qualche codice Morse o Braille. Non è nemmeno un semplice alfabeto manuale, ma una lingua con proprie regole, con proprie

forse con l'incapacità di far sì che la Commissione bilancio lavorasse al meglio, nel senso che quando si fanno le nozze con i fichi secchi diventa sempre tutto più difficile; ma abbiamo

la possibilità di interagire in modo serio con un mondo che a volte diventa una campana di vetro e non dà la possibilità di vivere serenamente.

Negli ultimi mesi, più volte, quest'Assemblea ha affrontato tematiche legate alla disabilità. Penso agli impegni che sono stati presi con le mozioni per le persone affette da sindrome di Down, e penso soprattutto alla legge cosiddetta del dopo di noi. Anche recentemente ho partecipato a tante iniziative sul mio territorio promosse da realtà che si occupano di disabilità e di inclusione: all'inaugurazione della nuova sede della sezione di Trento dell'Ente nazionale sordi piuttosto che all'assemblea di Anffas e a quella dell'Unione al Mart di Rovereto, il museo di arte moderna e contemporanea, si è tenuto il Mart *open day* con la presentazione di una video guida per non udenti realizzata nel linguaggio dei segni. Si tratta di un progetto che, da una parte, conferma l'attenzione da parte del museo di Rovereto nel favorire la fruizione artistica; dall'altra, è anche la dimostrazione che molti ostacoli possono essere superati. Inoltre, sempre al Mart, sono in corso altre sperimentazioni, che il Ministero dovrebbe favorire e guardare con grande attenzione, anche per applicazioni in grado di rendere i musei accessibili a tutti. Ho voluto menzionare queste realtà per dire come in ciascuna di queste circostanze ho potuto apprezzare i risultati e i tanti passi in avanti che sono stati compiuti per garantire una migliore qualità della vita, una migliore forma assistenziale ai disabili e alle loro famiglie, ma soprattutto per aumentare il grado di accessibilità alla vita comunitaria. Certo - l'ho già detto in quest'Assemblea - c'è ancora tanto da fare per rimuovere tutte le barriere materiali e culturali che ancora esistono. In Italia siamo spesso all'avanguardia per quanto riguarda i principi e le enunciazioni, ma troppo spesso siamo carenti sul piano dell'attuazione dei diritti. La lingua dei segni per sordi, sordociechi e disabili uditivi è una vera e propria lingua,

dopo la Convenzione ONU di New York del 2006, ratificata dal nostro Paese nel 2009. Il riconoscimento della lingua è essenziale per garantire a tutti il pieno accesso al sacrosanto diritto di ciascuno di potersi esprimere nella propria lingua. Sappiamo bene che si tratta non solo di un fatto simbolico, ma anche di un diritto sostanziale, che non può più essere rimandato nel tempo. In televisione, come nei grandi eventi pubblici, l'interprete LIS è sempre più presente, a riprova di una sensibilità sociale cresciuta nel tempo,

È assolutamente positivo che si sia giunti a un testo unitario, a dimostrazione che questo è un tema su cui le forze politiche devono trovare la convergenza. Molto importante è il lavoro che è stato fatto in Commissione e ne va dato atto a tutti i suoi componenti, ai presentatori delle proposte di legge, a tutte le colleghe e i colleghi che hanno lavorato sul provvedimento, ma soprattutto al relatore Russo che, grazie anche a una forte sensibilità, ha saputo fare una sintesi virtuosa di tutte le istanze emerse. È stato un lavoro di grande impegno, che ha coinvolto molte associazioni e realtà operanti nel settore e che ne ha raccolto le testimonianze, le richieste e il prezioso contributo d'esperienza. Voglio ringraziare, in particolare, l'Ente nazionale sordi e tutte le realtà che hanno collaborato, anche con me, e garantiscono sul territorio la possibilità per i non udenti di condurre una vita migliore, esprimere le potenzialità e valorizzare le competenze, l'impegno e il talento. Non ho dubbio nel dire che senza di loro, senza queste realtà preparate e motivate, oggi la nostra società potrebbe garantire ben poco. Dico questo con cognizione di causa, avendo seguito da vicino la preziosa e competente attività della sezione di Trento dell'Ente nazionale sordi. Il risultato di questo lavoro è nella completezza del provvedimento, che affronta davvero una pluralità di questioni tutte importanti. Per ragioni di tempo, vado per titoli: la prevenzione e l'identificazione precoce di fenomeni di sordità; gli interventi di sostegno psicologico; la costituzione di centri specializzati; l'aumento dell'accessibilità attraverso le nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* e *hardware* dedicati;

auspicio è che, una volta approvato il testo, si faccia in fretta con i decreti attuativi, ma soprattutto che si trovino le risorse indispensabili, non previste nel provvedimento in esame, per garantire effettivamente un diritto che è sacrosanto e sancito dalla Costituzione.

Per troppi anni alle persone affette da disabilità uditiva è stato negato il pieno diritto di cittadinanza e il provvedimento in esame è un importante passo per colmare finalmente questo colpevole ritardo.

Signor Presidente, vorrei innanzitutto ribadire che la sordità è una disabilità sensoriale e che pertanto va trattata con un adeguato protocollo sanitario: *screening* audiologico neonatale, diagnosi precoce, adeguata e tempestiva protesizzazione e abilitazione logopedica. La lingua italiana dei segni non ha più senso di esistere in istituti per sordi, tuttavia non si capisce come mai si continuano a finanziare. Già questa estate, attraverso il decreto-legge per il Mezzogiorno, è stato garantito un finanziamento per un milione di euro per il funzionamento degli istituti atipici e il corretto sviluppo dei processi cognitivi dei bambini sordi (così è scritto nell'emendamento),

Palermo, che è stato trasformato in un centro educativo diurno con assistenza scolastica e nulla ha a che fare con la didattica. L'istituto statale per sordi che ha sede qui a Roma ha esaurito dal 1° settembre del 2000, cioè anni fa, la sua attività scolastica in senso stretto; da tempo non riceve fondi pubblici e rischia di chiudere. Dopo anni di commissariamento sembra che ormai la sua fine sia segnata. Tutto questo per ribadire che questo disegno di legge, benché abbia avuto diverse e numerose modifiche, continua a essere, alla luce dei nuovi subemendamenti presentati dal relatore, una mera indicazione sulle possibili azioni che il Governo dovrebbe fare; indicazioni e consigli di programma, che nulla hanno a che fare con un reale impegno a garantire inclusione o eliminazione di ogni tipo di barriera che possa impedire alla persona sorda o sordocieca di poter agire, studiare, lavorare, in una parola vivere autonomamente, senza doversi sentire diversa o disabile perché non riesce ad accedere ai servizi che gli competono di diritto. Si continua ad incorrere nell'errore di considerare la sordità come uno *status* differenziato, quasi da proteggere, e non una disabilità da affrontare con un adeguato protocollo sanitario e logopedico, finendo così, inevitabilmente, non a offrire tutele ai soggetti che presentano tale disabilità, ma ad assicurare la permanenza dello stesso fattore diversificante. Le risorse economiche non sufficienti, tuttavia, creano i presupposti affinché siano sempre meno garantiti i diritti primari del cittadino, come il diritto alla salute e, in questo specifico caso, il diritto a una diagnosi precoce, alle protesi acustiche, alla riabilitazione, al sostegno scolastico e all'inserimento nel mondo del lavoro

e soprattutto la natura di tale problematica avrebbero dovuto suggerire che il lavoro si dovesse basare sul concetto più appropriato di inclusione più che sul concetto di integrazione. I bambini con gravi problemi uditivi fin dalla nascita sono solo lo 0,01 per mille dei cittadini italiani e oltre il 90 per cento di questi bambini con disabilità uditiva nascono da genitori udenti. Questo significa che, se si riuscissero ad approntare in modo corretto tutti gli interventi necessari che scientificamente oggi sono possibili e disponibili e se si intervenisse si intervenisse in modo celere con lo *screening* uditivo alla nascita, con la protesizzazione e con l'impianto cocleare, con la logopedia e con tutti gli strumenti tecnici a disposizione, il bambino con problemi uditivi, se ben supportato, potrebbe agevolmente raggiunge competenze linguistiche equiparabili a quelle delle persone senza problemi uditivi. La vera sfida dunque è proprio questa, ovvero quella di ottimizzare al massimo le risorse e di garantire percorsi efficienti e tempestivi. Per queste ragioni, al fine di garantire il pieno ed effettivo riconoscimento riconoscimento delle esigenze delle persone con disabilità uditiva e quindi al fine di riconoscere loro il pieno diritto all'inclusione sociale, sarebbe necessario che lo Stato non semplicemente promuovesse, ma garantisse un programma *standard* di iniziative e servizi in tutte le Regioni, per assicurare il diritto alla salute, alla parola e all'attivazione di processi virtuosi per garantire e non solo genericamente promuovere una reale parità di opportunità. Occorrono piani nazionali unificati e standardizzati, articolati a livello regionale per garantire prestazioni e

XVII)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare l'attenzione non solo dei colleghi parlamentari, ma anche del relatore e del Governo, su quelli che a mio parere rimangono nodi irrisolti del disegno di legge

che contraddistinguono il tentativo di garantire diritti in ordine a queste patologie e che potremmo fondamentalmente riassumere in due capisaldi:

e che confluiscono anche in uno strumento come la lingua dei segni e, dall'altra, i tentativi più recenti, legati anche alla tradizione oralista del nostro Paese, confluiti nell'adozione di nuove tecnologie che vanno normalmente sotto il nome di impianti cocleari. Queste due scuole di pensiero, se vogliamo definirle così, hanno provveduto nel tempo a giustificare misure che, nella visione del legislatore, a mio modo di vedere, devono essere tenute insieme con buonsenso ed equilibrio per poter fornire a tutti il rispetto non solo di un diritto, ma anche di una propria visione della realtà. È indubbio cioè che chi provvede a rimediare alla sordità tramite un impianto cocleare concepisce il male come privazione dell'essere. Per fare un esempio comprensibile, chi si ritrova per un incidente senza una gamba mira alla protesi, perché, attraverso quello strumento, colma un vuoto che è effettivamente ordinativo di una misura sociale, civile e di diritti ed è un tutt'uno con il rimedio alla patologia.

si pone sul livello educativo un problema molto serio: vi sono ragazzi, che sono stati impiantati già da bambini, che non vogliono imparare la lingua dei segni, ma intendono la possibilità di imparare la lingua italiana scritta e parlata (un tutt'uno questo profilo educativo) come la maniera più egregia di rispondere al proprio bisogno. bisogno. È vero o non è vero allora che introducendo questo nuova tipologia di intervento andiamo a creare una frattura all'interno della comunità italiana dei sordi? Se non fosse vero, probabilmente ci sarebbe già stata in questi ultimi decenni la possibilità di accordarsi in Parlamento. Si sarebbe trovato, nelle sei legislature che sono state descritte da chi è intervenuto prima di me, un possibile punto d'intesa. Nella realtà questo punto di intesa non lo si è trovato neanche in questa legislatura. Allora perché adottare questo provvedimento? il sospetto che questo provvedimento alla fine si risolva non tanto in qualcosa che trova rimedio al diritto dei sordi, quanto piuttosto in un provvedimento che trova rimedio all'esigenza degli interpreti della lingua dei segni di vedere riconosciuti i loro diritti e di vedere quindi previsto, all'interno del nostro sistema scolastico ed educativo, uno spazio che dovrebbe nel tempo, perché oggi non ha le risorse per farlo, trovare risposta ai loro bisogni. *(Applausi dei senatori da parte del relatore, una riflessione ulteriore, perché l'impostazione del provvedimento salvaguardi il diritto e la visione di tutti, il fatto cioè che migliaia e migliaia di famiglie hanno guardato all'introduzione delle nuove tecnologie in un modo che si lega con l'ordinamento dello Stato. È più agevole affrontare il problema della sordità con interventi risolutivi che sganciano la figura del sordo da quella di una persona assistita tutta la vita (tema dell'impianto cocleare) o è invece da preferire una sottolineatura che è anche culturale, che è insieme apertura ma anche chiusura alle ragioni del mondo di una piena integrazione? questi temi non per fare una polemica politica, consentitemelo. Da parte mia c'è semplicemente la volontà di mantenere insieme le ragioni di persone che, ferite dalla vita, possono invece trovare nel rapporto con le istituzioni piena accoglienza del proprio bisogno e dei propri diritti fondamentali. Mi auguro che il relatore, facendo ulteriori sforzi, come come sembra voglia enunciare anche attraverso alcuni suoi emendamenti, si ponga un problema ulteriore. Non rinuncio però a porre una questione che è ulteriormente dirimente. Questo provvedimento lascerà forse il Senato dopo questo voto per arrivare alla Camera, dove rischia di essere, ancora una volta, l'ennesimo provvedimento bandiera che non risolve una questione, ma che lascerà invece strascico nella prossima legislatura di tutto ciò che, sul piano del bilancio

Non nascondiamoci il fatto che questo provvedimento non è stato approvato nelle ultime sei legislature anche perché il mondo dei sordi italiani ha espresso posizioni molto diverse e la politica ha fatto fatica a trovare una sintesi di esse. Davvero vorrei che questo Parlamento, sia pure nelle sue ultime settimane, avesse invece l'ambizione di chiudere definitivamente questo percorso per aprirne un altro, perché questo testo non potrà essere risolutivo

proposito, anche rispondendo alle sollecitazione del collega Mario Mauro, tra gli emendamenti da me presentati ve ne è uno molto semplice, ma che reputo emblematico, che cambia il titolo di questo disegno

velo di dubbio dicendo che il disegno di legge in discussione vale per promuovere i diritti di cittadinanza di tutti i sordi italiani, nel pieno riconoscimento delle posizioni di ciascuno, come questo Parlamento deve fare. L'abbiamo detto più e più volte e lo ripeto ancora oggi:

ascoltando le richieste delle persone sorde del nostro Paese. È ad esse che noi dobbiamo rispondere oggi, al di là di ogni impostazione e di ogni visione che legittimamente, anche con un pizzico di ideologia, ci portiamo dietro rispetto a ciò che abbiamo ascoltato dentro

il percorso di rieducazione e riabilitazione può raggiungere risultati straordinari, quasi equiparabili a chi nasce con il dono straordinario dell'udito. Dobbiamo però essere franchi e dire che,

a chi ci chiede di riconoscere la lingua dei segni perché essa è lo strumento con il quale esercita la propria cittadinanza e il proprio modo di stare da protagonista nella società e nella propria comunità.

quale sia lo strumento attraverso il quale i sordi italiani possano e debbano esprimersi. Non è un diritto della politica decidere se la lingua dei segni o l'oralismo siano lo strumento attraverso il quale i sordi italiani possono esprimersi. Abbiamo sperimentato - e mi dispiace che alcuni di coloro che sono intervenuti non abbiano mai messo piede nella scuola di Cossato e in quella di Magarotto - e visto come i percorsi di bilinguismo siano oggi una punta avanzata dal punto di vista didattico e pedagogico. E lo dice un senatore che nella vita normale fa il docente di pedagogia. Quindi non si tratta di un ritorno al passato, di una ghettizzazione o della chiusura dentro l'idea del sordo come appartenente ad da proteggere e mantenere isolata. Devo dire infine che mi ha fatto male sentire quella che forse era soltanto una battuta della collega Rizzotti: immaginare, senza aver incontrato quei ragazzi, che insegnare nelle stesse classi, a bambini normodotati e a bambini non udenti, la LIS e la lingua italiana, contemporaneamente, sia come dare delle stampelle a dei bambini che possono camminare normalmente, significa davvero mancare di sensibilità, perché chi ha incontrato quei bambini, anche i bambini normodotati, sa quale straordinario valore pedagogico ha avuto per loro fare anche soltanto un gesto di avvicinamento nei confronti dei loro compagni meno fortunati

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare è il frutto di un lungo lavoro, che ha visto impegnati diversi Gruppi parlamentari, nell'intento comune di pervenire ad un testo unificato, consapevoli dell'esigenza di fare presto, visto che il nostro Paese è tra gli ultimi in Europa ad adottare una legge su questo tema. Come è stato già illustrato dal relatore, il senatore Russo, che ringrazio di cuore, il provvedimento in esame è volto a riconoscere i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, al fine di abbattere le barriere della comunicazione e della comprensione, promuovendo l'accessibilità agli strumenti e ai servizi finalizzati alla partecipazione e all'inclusione sociale, educativa, formativa e lavorativa:

Voglio sottolineare che, durante le numerose audizioni tenute in Commissione, si è potuto registrare un apprezzamento generale per l'iniziativa parlamentare, pur in presenza di divergenze, utili nel contraddittorio. Il testo oggi in esame ha recepito infatti alcune delle osservazioni emerse in quella sede, a conferma della positività del confronto. Al provvedimento di natura parlamentare il Governo ha dato il proprio convinto apporto, durante tutto l'*iter*, consapevole dell'urgenza di fornire delle risposte. Si tratta di temi che, personalmente, mi toccano moltissimo. Prima di concludere, un altro aspetto che mi preme evidenziare è che il disegno di legge in esame prevede l'intervento da parte di diverse amministrazioni, a vario titolo coinvolte, a testimonianza della finalità di costruire un tessuto quanto più omogeneo, sul quale poter innestare le misure necessarie

limitatamente alla parte relativa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché i subemendamenti 1.300/2, 1.301/1, 1.301/5, 3.300/1, 3.300/2 e 5.300/6, in quanto diretti a modificare il testo del disegno di legge e non l'emendamento al quale si riferiscono.

vorrei illustrare l'emendamento 1.101.

n. 104 del 1992 garantisce e certamente la differenza è notevole, perché garantire significa assicurare un impegno e un sostegno economico; promuovere è una buonissima intenzione che rimane nell'aria.

«tutte le forme di comunicazione alternativa aumentativa». Così, è importante curare l'acustica ambientale nelle scuole, al cinema, negli uffici, nei musei, nei tribunali per tutte le persone e gli studenti protesizzati. Ad esempio, in Inghilterra vi è un sistema di infrarossi e onde elettromagnetiche, proprio perché le persone portatrici di protesi non siano costrette ad aumentare il volume, con con un certo disagio della loro protesi, per poter eliminare il rumore di fondo. Quello che chiedono le persone protesizzate è avere il *wi-fi* che abbiamo normalmente e che dovrebbe esserci sempre, neanche a un grande costo. 1.106 recita: «La Repubblica adotta misure atte a garantire per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta».

incoscientemente sceglie per il proprio bambino la lingua dei segni anziché i metodi di comunicazione alternativa che lo facciano sentire normale? E questo glielo devo lasciar fare nel 2017? Non credo. *(Applausi del senatore

vi sono progetti come il telefono amplificato per i sordociechi o il progetto Parloma. Tutte queste forme alternative di comunicazione dovrebbero essere tutelate esattamente come il riconoscimento della lingua dei segni.

a scuola, ufficio, tribunale, RAI, università e per l'inserimento scolastico e lavorativo. intende ribadire cose già garantite: l'interprete lo può avere chi lo desidera, ma chi non lo vuole, ad esempio il disabile protesizzato, ha diritto all'assistenza, come ad esempio il miglioramento dell'acustica. PRESIDENTE.

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento da noi presentato, che interviene sull'affermazione di principio contenuta nell'articolo 6, solo che 6, solo che mette sullo stesso piano le varie tecniche che possono facilitare la comunicazione per le persone con delle difficoltà uditive. Ciò che noi rileviamo in questo disegno di legge è proprio il fatto che

(ma anche l'articolo 6), prevede che tutti gli interventi vengano fatti nell'ambito delle risorse già stanziate. Ebbene, nell'ambito di tali risorse (ed è la tesi che abbiamo portato avanti durante tutta la discussione), sarebbe augurabile avere una promozione dei vari tipi di intervento, non soltanto della lingua dei segni, ma anche degli altri metodi alternativi di comunicazione, come la lettura labiale e soprattutto la diagnosi precoce e gli impianti cocleari. Questo è quanto

Ma non è questo il principio con cui si dovrebbe agire. Noi riteniamo che gli interventi a favore delle persone con difficoltà uditive andrebbero adottati

agli impianti cocleari, che consentono una sensazione pari a quella di coloro che invece non hanno questi problemi. Pertanto, come si fa a mettere da parte questo e a privilegiare un solo settore? Benissimo, non abbiamo nulla contro la lingua dei segni, ma non può essere questa l'unica strada. strada. Ciascuno di noi conosce tantissime persone che non hanno intrapreso questa strada; nel caso di alcune persone non sapevamo neppure che avevano difficoltà uditive, perché comunicano esattamente come facciamo noi. questo è il punto ed è la ragione della nostra astensione su questo articolo, del nostro voto a favore dell'emendamento che stiamo per votare e della nostra astensione in generale su questo provvedimento.

Non costerebbe niente scriverlo, sarebbe uno stimolo alle Regioni per intervenire in questo senso, ma evidentemente le intenzioni del presente disegno di legge sono sono prevalentemente altre. Sono sicuramente buone, ma vanno soprattutto verso certi operatori, cui va tutto il rispetto, ma che

filiera di persone che svolgono un'importantissima opera di supporto, e cioè gli interpreti e gli insegnanti della lingua italiana dei segni.

l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, rimuovendo le barriere alla comprensione e alla comunicazione, non può che apparire un fatto positivo. Quello che occorre però fin dal principio sottolineare, colleghi, è il fatto che l'utilizzo della lingua dei segni non ci appare l'unico mezzo, e neppure la via migliore, per raggiungere questo scopo. L'utilizzo e il riconoscimento della LIS non esaurisce tutti gli strumenti possibili già oggi messi a disposizione dalla ricerca medico-scientifica. Di ciò si è dibattuto a lungo in Commissione nel corso delle numerose audizioni che si sono svolte con esperti del settore e rappresentanti di associazioni. Il provvedimento in esame, come detto, si propone di garantire diritti e tutele ai soli cittadini sordi con disabilità uditiva in genere e ai sordociechi. Nulla di più nobile, se non fosse che questa parità di diritti ci risulta essere già pienamente presente nell'attuale ordinamento italiano. Al fine di ottenere questi risultati, si richiede la rimozione delle barriere che si frappongono alla comprensione e alla comunicazione, la rimozione cioè di tutti i potenziali ostacoli al pieno sviluppo della persona, all'effettiva partecipazione alla vita collettiva e all'accesso all'informazione. Sono quindi previste, dal testo legislativo all'esame dell'Assemblea, diverse forme di promozione dei sistemi di sottotitolazione, dei servizi di interpretariato in lingua dei segni e in lingua dei segni tattile e iniziative di promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico. Colleghi, proprio perché sposiamo completamente la volontà di rimuovere le barriere, che ancora oggi impediscono la piena partecipazione dei cittadini con disabilità uditive, sordi e sordociechi e proprio perché vogliamo unirci agli sforzi utili per supportare iniziative realmente utili, non possiamo che manifestare tutti i nostri dubbi sull'efficacia delle misure previste in questo testo. Non siamo certi cha la promozione di una lingua dei segni e la spinta per la sua diffusione costituiscano la strada giusta da seguire. Pensiamo invece che l'integrazione delle persone affette da una tale disabilità possa e debba avvenire piuttosto tramite la logopedia,

alla ricerca scientifica in questo campo. I nostri dubbi si fanno ancor più seri se valutiamo le proposte in essere che riguardano l'ambito scolastico. L'età educativa, infatti, riguarda una fase della vita particolarmente importante per lo sviluppo di competenze in grado di abbattere le differenze comunicative. Il provvedimento dispone che siano garantiti nelle scuole la figura dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni sordociechi, oltre alla figura dell'interprete in LIS e LIS tattile. Nell'ambito universitario e postuniversitario si ricorre alla stenotipia, al respeakeraggio, oltre che alla lingua italiana dei segni e alla lingua italiana dei segni tattile. Proprio in merito al settore dell'educazione riscontriamo criticità rilevanti che, a tutela e a protezione dei più deboli, non possiamo che sollevare con forza in questa sede. Il disegno realizzato per garantire l'inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche ha utilizzato una tavolozza di colori parziale, per non dire monocolore, riservando un ruolo di esclusività alla lingua italiana dei segni quale strumento per ottenere la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione. Ebbene, colleghi, la lingua dei segni ha sì una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale, ma mai potrà sostituire completamente la lingua italiana. In essa è infatti assente la forma scritta. Inoltre - fatto molto importante - la LIS non può esprimere un linguaggio metacognitivo, quindi garantisce minori possibilità affinché si possano realizzare in tutti gli studenti, anche quelli con difficoltà, apprendimenti significativi, accompagnati da un incremento di capacità a livello cognitivo. Ciò è dimostrato banalmente anche dal fatto che la lingua dei segni deve essere continuamente integrata dall'italiano scritto, dalla dattilogia, dalla lettura labiale propria della lingua parlata, ad esempio per esprimere termini scientifici o astratti, nomi propri, di luogo e molto altro. Come detto, incentrare tutta l'attenzione di noi legislatori, tutti gli sforzi e tutte le risorse sulla lingua dei segni ci appare di per sé un grave limite. Anzi, ci fa pensare, colleghi, che il provvedimento in esame non sia scaturito da intenzioni nobili, bensì da altre motivazioni. Come mai nel provvedimento non è stato previsto alcun intervento di sostegno alla logopedia, metodologia considerata fondamentale dalla scienza medica, per realizzare processi abilitatiti e riabilitativi? Come mai non si prendono in considerazione tecniche alternative come quelle di riabilitazione alla parola? Perché non si mettono i genitori in condizione di poter scegliere liberamente il tipo di riabilitazione ed educazione cui sottoporre il figlio? Colleghi, gli obiettivi che ci siamo posti di inclusione sociale, accessibilità totale, rimozione delle barriere, facilitazione della comprensione e della comunicazione non possono essere raggiunti se non siamo onesti e realisti con noi stessi. Un percorso di riabilitazione deve tenere conto della realtà, cioè del fatto che la maggior parte dei cittadini non conosce la lingua dei segni e che, quindi, se ad un bambino è stata insegnata solo questa modalità di comunicazione, questo bambino, raggiunta l'età adulta, si troverà a dover affrontare una condizione di inevitabile e drammatico isolamento nel momento in cui dovrà affrontare il mondo del lavoro e la vita sociale. Ecco perché ci permettiamo di rilevare in questa sede che la scelta di incentrare gli interventi in modo prioritario e quasi esclusivo sull'uso della lingua dei segni potrebbe rappresentare un grave e imperdonabile errore di valutazione. Per questo motivo, pur condividendo l'intento di questo provvedimento e riconoscendo l'importanza del tema trattato, riteniamo di dover esprimere un voto di astensione, nella speranza che questo segnale possa essere colto come occasione per rimodulare gli interventi in cantiere.

Questo è probabilmente certo. Si potevano mettere più soldi? Probabilmente era necessario. Alla domanda se, poi, questo sia l'unico metodo valido per affrontare tale problematica abbiamo già abbondantemente risposto di no, ma è sicuramente un buon inizio. L'idea di portare avanti un provvedimento di questo tipo nasce sicuramente della necessità, come abbiamo detto anche in discussione generale, di mettere in condizione 960.000 persone persone - ragazzi, giovani o meno giovani - che hanno difficoltà nell'inserimento all'interno della società e ad avere rapporti

in modo serio con i coetanei; non meno importante è la questione dell'inclusione lavorativa. A volte ci si dimentica della problematica della formazione permanente che questi ragazzi, portatori di una

alle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, quali punti in cui sia previsto un servizio di interpretariato in LIS. Sono tutte attenzioni che

che fortunatamente non è avvenuta. Tenendo la barra dritta, il relatore, per quanto mi riguarda, ha fatto un buon lavoro e siamo potuti arrivare a una votazione

Presidente, non aggiungo altro e dico semplicemente che il Gruppo della Lega voterà favorevolmente sul provvedimento in esame, nella speranza che esso venga affinato, magari nel prosieguo

con disabilità che detta la cornice su cui legiferare in merito alla tutela dell'identità culturale e linguistica delle persone sorde. In particolare, secondo l'articolo 21, della stessa gli Stati devono provvedere ad accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni e a riconoscere e promuovere l'uso di tale lingua. La ratifica della Convenzione ONU da parte del nostro Paese vincola dunque il legislatore a emanare una normativa interna conforme ai diritti e ai nuovi *standard* di tutela in essa stabiliti. Finalmente lo stiamo facendo. Ho parlato di legge controversa anche perché siamo di fronte a una regolamentazione normativa attuale molto frammentata, che direttamente o indirettamente si occupa anche della sordità e delle sue implicazioni. Non si è ancora potuta superare una produzione normativa così disomogenea a causa di un dibattito caratterizzato da posizioni culturali diverse, come quelle di coloro che rifiutano categoricamente il riconoscimento della lingua dei segni italiana ritenendola una mera tecnica di supporto o un linguaggio mimico-gestuale, oppure auspicano un riconoscimento senza però voler accordare tutela agli aspetti dell'identità culturale e linguistica o, infine, reclamano con forza un riconoscimento della LIS come lingua minoritaria. Una posizione, questa, che ho sostenuto non solo alla luce della ratifica italiana della Convenzione ONU, ma soprattutto in nome del diritto fondamentale di ognuno ad esprimere se stesso nella propria lingua - vocale o visivo-gestuale che sia - e a identificarsi con essa. Credo sia giusto ricordare, a questo proposito, che la stessa comunità dei non udenti si è divisa tra sostenitori della lingua dei segni come lingua naturale per i sordi e coloro invece che mirano a progressi medici e all'apprendimento della lingua parlata grazie ad ausili tecnologici. La sordità è un *handicap* non immediatamente riconoscibile, ma comporta implicazioni negative in tutte le attività sociali della persona, dell'accesso all'informazione, ai servizi, al lavoro, alle prestazioni assistenziali e sanitarie siamo ancora, purtroppo, molto in ritardo, perché restano troppi impedimenti quali la carenza di figure professionali specializzate, di attrezzature tecniche specifiche, di servizi telefonici "ponte" e di SMS per le emergenze. è, insomma l'esigenza primaria per il legislatore di favorire l'inserimento dei sordi nella vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva e intellettuale, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le amministrazioni dello Stato. Insomma: il riconoscimento della lingua italiana dei segni può diventare davvero un progetto di vita per i sordi, cittadini che non sono pienamente integrati perché hanno il problema oggettivo di non poter interloquire con chi non conosce la lingua dei segni. Tutte le associazioni e le famiglie audite in 1a Commissione ci hanno detto di fare presto una legge che riconosca ufficialmente la lingua dei segni anche in Italia, ultimo Paese in Europa a dover fare ancora questo passo.

e la promozione dell'autonomia degli individui, oltre alla facilitazione del processo di integrazione delle persone sorde nella società moderna. Occorre tener conto anche di un altro elemento importante, ossia che la lingua dei segni permette il superamento delle difficoltà comunicative legate anche ad altri gravi *handicap* come l'autismo. Nel corso delle audizioni, abbiamo anche appreso che non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino che la lingua dei segni costituisca un ostacolo nell'apprendimento della lingua parlata. Dunque, entrando nel merito della legge che siamo chiamati ad approvare, la domanda da farsi è se risponda pienamente alla Convenzione ONU e se, soprattutto, vada concretamente incontro alle richieste della comunità interessata. Dal punto di vista dei principi, non c'è dubbio che questa sia una buona legge, perché formula i diritti delle persone sorde e la rimozione delle barriere della comunicazione attraverso tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, riconosce alle persone sorde la libertà di scelta sulle modalità di comunicazione, prevede interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi, prevede l'accessibilità universale di ambienti, beni, processi, servizi e dispositivi, chiede alla pubblica amministrazione di garantire la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno con la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, con l'estensione di queste garanzie anche al percorso universitario e post-universitario. Una delle due principali novità introdotte, infine, è l'istituzione presso il MIUR del Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei segni italiana e l'altra è l'istituzione al Ministero del lavoro dell'Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità, in rappresentanza delle principali associazioni. Tutto bene, dunque? Dopo l'articolo 13, che affida al Governo il compito di monitorare l'attuazione della legge e predisporre le sanzioni per le violazioni, l'ultimo articolo, che riguarda l'invarianza finanziaria, precisa

Mi chiedo in conclusione, dando atto al relatore Russo del grande lavoro di mediazione svolto ed annunciando il nostro voto favorevole, se le buone intenzioni di questo disegno di legge non finiranno per scontrarsi con l'amara realtà della mancanza totale di risorse. Speriamo davvero di no, perché sarebbe una beffa. *(Applausi della mi piace iniziare questo mio intervento in dichiarazione di voto a nome del Gruppo delle Grandi Autonomie e Libertà sottolineando l'impegno morale che è già contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge: «la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione

straordinaria perché va ripreso il contatto con le fasce più deboli del Paese ed il Parlamento non può che trovare un'occasione favorevole, come in questa giornata, nell'approvare con una larghissima maggioranza un provvedimento che tornerà utile, quantomeno, a segnare cammini di civiltà per quanto riguarda l'*handicap* uditivo e visivo. Mi sembra utile, tra l'altro, anche sottolineare, ancora al comma secondo dell'articolo 1, che «la Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio»

vi sia un po' tutto il senso della legge, specialmente quando si parla di arte, cultura, tempo libero e trasporti dedicati alle persone portatrici di questo *handicap*. Mi sembra che le visite guidate nella lingua italiana dei segni, le videoguide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, le applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura ed al tempo libero libero siano fattori da mettere in evidenza e da sottolineare con grande positività. Lo stesso dicasi per quello che è previsto per il settore dei trasporti, che sappiamo essere il lato debole, il vero *handicap* per chi è affetto da queste infermità, ovvero la

funzionamento dei trasporti pubblici e la sicurezza nei trasporti pubblici, specialmente per quanto riguarda le emergenze, che devono essere comunicate attraverso la LIS e sottotitolate. Presidente, mi sembra che in questo campo l'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione nella lotta dell'umanità contro le disabilità uditive e visive può riconciliare insperatamente Internet,

la scienza, la tecnica e la tecnologia possono esplicare i loro benefici per l'umanità intera. Ahimè, non sono granché le disponibilità e le risorse che in generale corroborano e connotano questo disegno di legge, e qui noi chiediamo un ulteriore sforzo al Governo affinché ponga mano al portafogli e metta a

Il disegno di legge infatti intende abbattere barriere ed ostacoli all'integrazione, che sono attualmente di natura fisica, psicologica, morale e culturale.

nella lingua dei segni. Quando abbiamo avuto le immagini sotto i nostri occhi, tutti siamo rimasti stupiti dall'efficienza: quasi un senso di straniamento. È un altro mondo e questo mondo deve essere assolutamente elaborato e percepito anche dalle persone che non hanno questo *handicap*. Altrettanto straordinario è il ricordo del film «Lezioni di piano» della regista australiana Jane Campion, che ci dice quanto sia straordinario quel mondo fatto di silenzi, ma anche di profonde emozioni. Con questi sentimenti, dichiaro il voto favorevole

sopra il Gruppo Art. 1-MDP voterà a favore di questo provvedimento, perché dopo tante discussioni, rinvii e ordini del giorno, è necessario mettere un punto fermo e fare qualcosa di concreto per tutelare i diritti delle persone con disabilità uditive in genere e delle persone sordocieche,

per cercare di armonizzare le diverse correnti di pensiero che sono state oggetto di un approfondito dibattito e di accesa discussione. Mentre apprezziamo il fatto che si sia evitato nel testo il richiamo all'articolo 6 della Costituzione o all'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che avrebbero indotto a inquadrare le persone sorde come minoranza linguistica o come comunità di diversi, ci sembra ancora sbilanciata l'attenzione sulla LIS o sulla LIS tattile. Apprezziamo il fatto che nell'articolo 3 si preveda la promozione dell'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, come le indagini preventive in gravidanze, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica anche al fine degli appropriati interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce,

Voteremo comunque a favore perché soprattutto il provvedimento prevede la libertà di scelta delle persone sorde e delle loro famiglie circa le modalità di comunicazione, i percorsi educativi e gli ausili da utilizzare per raggiungere il pieno sviluppo della persona e la sua piena inclusione sociale. Voteremo a favore perché nel testo si parla finalmente di inclusione e non più di integrazione, superando un modello focalizzato solo sul *deficit* della persona e rispettando i principi di non discriminazione, di pari opportunità, autonomia e indipendenza. Evito di

È iscritto a parlare il senatore Panizza.

il passaggio che questo disegno di legge finalmente compie verso l'inclusione di gruppi comunque svantaggiati rispetto a una maggioranza di consociati, per cui non si può che essere favorevoli a un'iniziativa di questo genere. Il tema è tipico della tutela delle minoranze perché il problema non è tanto la definizione di chi faccia parte di minoranze; non c'è nulla di più congiunturale, di più occasionale dell'essere minoranza: tutti possono trovarsi in posizioni minoritarie, a seconda del contesto e del momento. Non si tratta solo di minoranze etnico-linguistiche, religiose, culturali, ma anche, per l'appunto, di minoranze come quelle di cui stiamo parlando in questo momento con riferimento alla caratteristica dell'espressione, e quindi dell'inclusione all'interno della società. Per questo è importante non tanto soffermarsi sulle definizioni, su chi faccia parte di una determinata minoranza e su come si possano definire i gruppi, quanto, soprattutto nell'ottica del legislatore, stabilire gli strumenti. ad approvare mette a disposizione finalmente strumenti per i quali le persone sorde hanno atteso fin troppo tempo. Certo, ci sono state molte discussioni rispetto alla validità dello strumento: le ha ricordate molto bene il relatore, quindi non mi soffermo. Il punto è che senza gli strumenti sappiamo che si ha esclusione; con lo strumento si può dare inclusione, e se ci fossero accorgimenti da prendere, modifiche da fare, il legislatore dovrà essere pronto a testare l'efficacia l'efficacia normativa del provvedimento sul medio e lungo termine. È essenziale prevedere la cornice giuridica entro la quale colmare il *deficit* di inclusione che un determinato gruppo, particolarmente svantaggiato in determinati contesti, non soltanto quello di Per questo, finalmente, la previsione dello strumento, nonostante le seppur interessanti obiezioni che sono venute in questo dibattito e nei dibattiti precedenti - sappiamo che questo strumento arriva in ritardo - potrà potrà sicuramente essere utile, ma lo si dovrà testare *ex post*. Quindi, è importante innanzi tutto aprire la strada al provvedimento e poi essere altrettanto umili e disponibili quando si tratterà eventualmente di modificarlo, qualora ciò si renda necessario. Per i motivi esposti, il voto

Premetto tutto questo perché è chiaro che senza risorse, non esiste alcun diritto di cittadinanza e inclusione. Giusto per chiarire a chi ci ascolta,

il trasporto degli alunni con disabilità per l'anno scolastico. La preoccupazione è ancor più inaccettabile perché mancano le risorse proprio per garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità.

emendamenti per finanziare lo *screening* uditivo alla nascita, ogni intervento diagnostico precoce, un corretto protocollo sanitario per la protesizzazione, l'impianto cocleare, la logopedia, l'aiuto della tecnologia da garantire in tutte le Regioni, con lo stesso *standard*

lo *screening* uditivo. È vero, ciò spetta alle Regioni, ma è chiaro che non c'è un diritto di opportunità garantito a tutti, perché non in tutte le Regioni viene fatto. Il disegno di legge in esame ha confrontato visioni diverse, cercando in parte di tenerle insieme. Tuttavia, per quanto ci riguarda, il risultato è un coacervo di norme che non tengono conto di cosa è accaduto negli ultimi anni e degli importanti cambiamenti culturali e sociali dovuti anche all'utilizzo di importanti nuove tecnologie. Se parliamo di diritti di cittadinanza, vuol dire che parliamo di uguaglianza, di inclusione e di piena attuazione di quel grande manifesto dell'uguaglianza che è proprio l'articolo 3 della nostra Costituzione, quell'articolo che ci consente di parlare di disabilità e di persone sorde oltre gli stereotipi e i luoghi comuni. Non è possibile considerare le persone sorde come una minoranza linguistica, perché paradossalmente sarebbe altissimo il rischio di ghettizzazione. Ci preoccupa molto, ad esempio, l'articolo 5 sull'inclusione scolastica, perché proprio la mancanza la mancanza delle risorse e il rinvio alle amministrazioni locali (cioè quelle sottoposte ai tagli più feroci sul *welfare*) per garantire l'inclusione scolastica è davvero un paradosso. Non troviamo traccia nella legge di assunzione di insegnanti di sostegno e di assistenti scolastici. La scuola è iniziata da pochissimo e tutti noi sappiamo che mancano gli insegnanti di sostegno, per non parlare degli assistenti alla comunicazione. Ad esempio nella mia città, a Firenze, abbiamo assistito addirittura a una guerra tra disabili, la cosiddetta guerra tra poveri, perché gli assistenti alla comunicazione, in mancanza di risorse dello Stato, vengono contesi tra più bambini. Il senatore Russo ci ha chiesto se noi abbiamo visitato le esperienze di eccellenza. Beh, io chiedo al senatore Russo se ultimamente ha

di fare attenzione a non istituzionalizzare solo questo percorso e a non limitare la possibilità dei disabili uditivi, al fine di garantire le tante opportunità. La sordità non è uguale per tutti: l'85-90 per cento dei nati sordi nasce da genitori udenti e molti sordi lo sono diventati

può essere di aiuto a superare i limiti di questa legge, soprattutto nella fase attuativa. Però - ripeto - il limite più grande di questa legge è l'assenza di risorse. Abbiamo ascoltato e abbiamo visto che l'articolo 9

le risorse delle Province autonome di Trento e Bolzano. Noi siamo contenti di questa grande esperienza al Mart, inaugurata pochi giorni fa, ma vorremmo che quella garanzia fosse assicurata in tutte le Regioni e a tutte le persone con disabilità uditiva. Questo rinviare ancora una volta alle Regioni e agli enti locali, è un po' come dire che abbiamo fatto una legge di principi e che poi vedremo cosa succederà. Insomma, avremmo voluto la garanzia del diritto di cittadinanza e non soltanto la sua promozione. I bambini che nasceranno sordi sordi potranno raggiungere una competenza linguistica al pari di quella degli udenti e i sordi non dovrebbero essere più costretti a gesticolare per farsi comprendere. Negli ultimi vent'anni sono stati fatti grandi progressi e, se ci fossero davvero le risorse, la scelta della LIS potrebbe rimanere un'esperienza limitata; questo avrebbe dovuto essere il vero obiettivo della legge. Ancora una volta, dopo tante parole, restano gli slogan; invece, con il coinvolgimento di ricercatori, professionalità associazioni, si sarebbe potuto contribuire a modernizzare l'applicazione di una legge che, per quanto ci riguarda, guarda indietro a trent'anni fa. Per tutte queste motivazioni, Sinistra Italiana si asterrà.

e che giunge qui in Parlamento comunque svuotato del suo senso principale, quello di creare inclusione ed evitare divisioni tra chi può permettersi impianti all'avanguardia e chi invece deve accontentarsi delle miopi e minuscole risorse regionali, quando ci sono. Si continua a incorrere nell'errore di considerare la sordità come uno *status* differenziato, quasi da proteggere, e non una disabilità da affrontare con adeguati protocolli sanitari. Abbiamo visto che nel testo del disegno di legge il Ministero della salute non viene nemmeno citato. citato. Succede quindi che le risorse economiche non sono sufficienti, non si creano i presupposti affinché siano veramente garantiti i diritti primari del cittadino, come il diritto alla salute, e tutto questo non fa altro che creare divisioni divisioni e differenziazioni, ma assolutamente non inclusioni. Ancora oggi lo *screening* audiologico neonatale è garantito, con protocolli non omogenei, in meno della metà delle Regioni italiane. In alcune Regioni la diagnosi di sordità viene effettuata dopo i due anni del I risultati nelle sordità preverbali, a parità di perdita uditiva, sono migliori quando è minimo il tempo intercorso tra il sorgere della perdita uditiva e il ripristino della sua funzione.

passare dal «promuovere» al «garantire. Specie quando si tratta di operare dentro le scuole, sul tema della professionalità degli insegnanti, perché non si pone un accento su corsi di laurea specifici?

La differenza che sussiste tra il concetto di promuovere e quello di garantire è che nel primo caso si è disponibili ad impegnarsi per raggiungere un risultato, mentre nel secondo semplicemente si assicura il raggiungimento del risultato. Questo provvedimento è certamente migliorato rispetto al testo iniziale e sono sicuramente apprezzabili gli sforzi e la direzione intrapresa. Tuttavia, crediamo che si sia persa un'occasione per intervenire in maniera decisa al fine di affrontare al meglio i problemi delle persone con disabilità uditiva. L'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire, anche al non udente - qualsiasi non udente, in qualsiasi città di questo Paese - il proprio ruolo di cittadino,

Non deve essere la persona sorda a preoccuparsi di intraprendere dei percorsi che gli consentano di essere incluso, ma deve essere lo Stato a garantire l'inclusione reale. Per tutto questo il Gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà dal voto.

chiedere a tutte le persone diversamente abili nel settore della sordità di capirsi, ma per fare questo bisogna parlarsi e per parlarsi bisogna ascoltarsi.

un'ingiustizia, una trascuratezza, una cosa grave. Voi pensate davvero che il Lussemburgo, che ha il reddito *pro capite* più alto di tutti i Paesi europei (100.000 euro annui a persona) non avesse voglia di riconoscere un diritto o che

Abbiamo addirittura la terapia genica sperimentale per la rinascita delle cellule ciliate, studi del Boston Children's Hospital, della Harvard medical school per restituire ad esempio l'udito nella sindrome di Usher, che è una malattia genetica rara, ma che proprio per questo dovrebbe essere riconosciuta precocemente.

tutelare e garantire (non promuovere) i diritti dei disabili, compresi quelli uditivi.

tutte le persone con disabilità uditiva possano intendersi in qualsiasi posto vadano, se non hanno avuto la possibilità di avere protesi sofisticate o impianti cocleari, che in Italia nei casi necessari vengono forniti dal

Non tutti forse in quest'Aula sono a conoscenza del fatto che una bambino con disabilità uditive non sarà mai veramente bilingue, perché ci sono due metodi con *feedback* diversi, visivo e uditivo. Se è più comodo il visivo, sarà per lui compromessa l'acquisizione della della lingua verbale e ridotta anche la capacità evolutiva, come dimostrano studi scientifici, le società scientifiche di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria. Spererei in un prossimo futuro dove non ci siano classi bilingui, ma bambini che non abbiano più bisogno della lingua dei segni. Un bambino che non abbia più bisogno dell'interprete. Già gli interpreti sono numerosi. Ho visto in Rete molte scuole di interpretariato per la LIS e, magari, pensare ad una reale formazione non sarebbe male.

ad esempio, con una formazione come insegnante di sostegno, come assistente alla comunicazione. È già stato ricordato come i *tutor* della cosiddetta buona scuola, non stiano riscuotendo molto successo, visti i ricorsi di genitori disperati. E sarebbe questo un altro argomento da approfondire.

Sarebbe fondamentale perseguire il diritto alla salute preventiva con piani nazionali e regionali e, come ho ricordato, la prevenzione in gravidanza di malattie infettive del sistema TORCH. diagnosi precoce in tutti i punti nascita in Italia entro i tre mesi di vita. Il Piano sanitario 2011-2013 lo indica come priorità, ma è attuato solo in una decina di Regioni. poi richiesta l'applicazione dei LEA per lo *screening* perinatale precoce; anche questo avviene a macchia di leopardo ed è gravissimo. Sarebbe inoltre meglio avere una precoce protesizzazione e non impianti tardivi. implementare i logopedisti, perché sono troppo pochi e in alcune Regioni quasi inesistenti; le famiglie sopportano costi proibitivi e spostamenti massacranti, percorrendo anche più di 100 chilometri, per far seguire privatamente i loro bambini. implementare i Centri regionali audiologici che, ad esempio, non esistono in Sardegna. Vi è bisogno di curare l'acustica ambientale nelle scuole, per gli studenti protesizzati, nei cinema, nei musei, negli uffici pubblici e nei tribunali. Tutto questo richiede risorse e, forse, i colleghi non ricordano che nella proposta di legge discussa in quest'Assemblea a maggio e a giugno, era previsto un fondo di due milioni di euro, finalizzati alla realizzazione dell'articolo 3.

quindi un'altra legge perfetta nell'intenzione, ma difficile nell'applicazione, come ad esempio la legge sull'autismo? O vogliamo parlare della legge sul dopo di noi? Cerchiamo di essere seri. Come Forza Italia abbiamo discusso del provvedimento

una quotidianità così dolorosa. Un Governo che trova cinque miliardi per fronteggiare il problema dell'immigrazione, non trova due milioni di euro, senza togliergli a qualcun'altro, per migliorare ed ampliare i diritti delle persone disabili uditivi.

garantisce e non promuove. E perché legiferare oltre se la persona sorda si integra nella scuola di tutti, parlando, leggendo e studiando come tutti? Perché non utilizzare queste risorse per potenziare la parola con i sottotitoli, ad esempio con l'insegnante di sostegno? Perché legiferare oltre se la LIS, per chi la vuole, è già contemplata dalla legge n. 104 del 1992? Per questi motivi Forza Italia si asterrà

il testo così proposto dalla 1a Commissione e, a mio parere, efficacemente emendato dall'Assemblea, a partire dal titolo, partire dal titolo, esprime e favorisce la piena attuazione di tre principi costituzionali fondamentali. Essi sono stati ampiamente richiamati nel ricco dibattito

il diritto alla piena inclusione sociale, il diritto alla rimozione di ogni forma di discriminazione, che possa ostacolare il raggiungimento della dignità della persona,

Quest'ultimo principio, onorevoli colleghi, include infatti in modo innovativo e per la prima volta con riferimento alle persone con disabilità uditive nella legislazione italiana il riferimento al diritto alla lingua, inteso nella sua accezione più moderna, più qualificante e più importante per capire il senso di questa

corredano la vita della nostra società - ha rappresentato un punto mancante, che finalmente viene colmato nella legislazione italiana. Lasciatemi dire dire e soffermarmi molto brevemente su questo punto, che è un passo decisivo, lungamente atteso soprattutto dalla comunità scientifica, che in Italia come in altri Paesi ha prodotto, nel corso degli anni, una vastità di studi e di ricerche di carattere teorico e metodologico, che finalmente potranno essere applicati al modello educativo bilingue tra lingua dei segni e lingua italiana. Il modello del bilinguismo potenzia in maniera inequivocabile - la scienza non lascia dubbi a tale riguardo, come in molti altri casi - la possibilità di recuperare, di valorizzare e di rendere effettivamente attuata la capacità cognitiva e comunicativa dei bambini con disabilità uditiva di vario genere. Gli studi sul bilinguismo - lingua dei segni e lingua, in questo caso, italiana

la plasticità percettiva, la capacità di adattamento a diversi contesti e soprattutto - lasciatemi dire, forse questo è il tratto determinante - lo sviluppo di una personalità più aperta, più flessibile e più incline all'adattamento alla dinamicità del contesto sociale, che è ciò che la società oggi chiede. È già stato detto, ma lo voglio ripetere, citando una tradizione di studi, soprattutto nel nostro Paese, assolutamente autorevole, che che la lingua dei segni è a tutti gli effetti strutturalmente una lingua, come quelle naturali. In questo senso, come ogni esperienza di bilinguismo, l'apprendimento di una seconda produce un vantaggio cognitivo, psicologico e sociale che è solo un arricchimento, fondamentale per l'esperienza dei bambini che si troveranno a poter usufruire anche di questa possibilità. Ho avuto l'opportunità - e vorrei ricordarlo, signor Presidente - da Ministro dell'istruzione di vedere concretamente, nelle classi della piccola scuola di Cossato, in Provincia di Biella, o del più celebre istituto Antonio Magarotto a Roma o anche in altri istituti che stanno sperimentalmente adottando questo modello (penso all'istituto comprensivo Giovanni Modugno di Barletta), l'efficacia, l'efficacia, non solo educativa, ma anche di progresso cognitivo che questo strumento può garantire ai bambini non udenti e a quelli udenti. Ciò che è stato detto anche da chi ha annunciato il proprio voto di astensione in Aula prima di me rappresenta un altro punto che è importante sottolineare e che vorrei ricordare ai colleghi, ossia il fatto che negli articoli 5 e 6 e nell'articolo 3, in particolare, questo disegno di legge tenga conto di tutti i risultati della ricerca scientifica, non solo degli studi di didattica e glottodidattica applicati al bilinguismo LIS-lingua italiana, ma anche e soprattutto dell'avanzamento nel campo della medicina preventiva (è stato ampiamente citato lo *screening* neonatale, l'indagine preventiva in gravidanza) e della medicina riabilitativa. Con questa legge l'implantologia cocleare diventa uno strumento, sicuramente già esistente nel Paese,

che la scienza e la politica oggi si ritrovino congiunte in un obiettivo di civiltà molto atteso nel Paese. Quella che ci ma lascia liberi di compiere una scelta fondamentale per l'avanzamento e il progresso, sia nella fase di apprendimento dei bambini, sia nella vita adulta di coloro che, purtroppo, sono affetti da questa disabilità, per nascita o per successive esperienze;

vuole semplicemente introdurre nuovi strumenti o nuove metodologie di aiuto alla condizione della sordità; un provvedimento che esprime semplicemente e crucialmente un'istanza di civiltà. E quando le leggi non impongono, ma lasciano lasciano libertà di scelta, quando esprimono un'istanza di civiltà sono buone leggi, devono essere votate positivamente e offerte alla società che è fuori da quest'Aula come un contributo che, in questo caso, beneficia dei risultati della scienza, ma li traduce efficacemente, anche se tardivamente, in un atto politico importante*.

che quando non si conosce un argomento si dovrebbe stare zitti o quantomeno, prima di parlare, sarebbe necessario informarsi, meglio se con le persone giuste. Infatti ci vuole sempre rispetto. Io, per esempio, non essendo medico, non mi sognerei neppure di dire ad un chirurgo come operare. Invece, quando si tratta di lavoro e di sindacato tutti diventano esperti, naturalmente con il sedere degli operai. L'ultimo in ordine cronologico, l'onorevole Di Maio (evidentemente Cernobbio fa brutti scherzi)

in primo luogo, pochi mesi fa, grazie al popolo italiano siamo riusciti a difendere la nostra Costituzione da un attacco senza precedenti. In ballo, se non sbaglio, c'erano appunto la democrazia, la rappresentanza e l'autonomia del Parlamento. Ora devo pensare o che l'onorevole Di Maio non sappia che il sindacato è un'associazione libera e democratica prevista dall'articolo 39 della nostra Costituzione

Il secondo punto grave è che l'onorevole Di Maio, essendo di Pomigliano d'Arco dove c'è una storia operaia importante, magari dovrebbe stare un pochino di più con i lavoratori e meno a Cernobbio, un posto che fa brutti scherzi a quanto vediamo. Magari avrebbe appreso cose importanti relativamente al lavoro e ai sindacalisti. Per esempio cosa rischiano i tanti lavoratori che fanno anche sindacato per passione, quella passione che serve per poter difendere la democrazia e la dignità nei luoghi di lavoro. Magari gli darebbero dei consigli relativamente a ciò che serve ai lavoratori per migliorare il sindacato, ma questo lo possono fare e lo devono fare solo i lavoratori, non deve Servirebbe una legge sulla rappresentanza, gli direbbero, perché ai lavoratori viene negata la possibilità anche di votare da chi farsi rappresentare e noi qui in Senato dovremmo essere ancora più convinti di questo. *(Il microfono si disattiva

Dovremmo fare una discussione molto più seria su quei disastri che ha provocato il *jobs act*, sugli amici di Cernobbio, perché qui sta il vero problema. qui sta il vero problema. Ormai, infatti, i lavoratori non possono più pretendere nemmeno la sicurezza sul lavoro, perché senza diritti non si può pretendere nemmeno questo.

Signor Presidente, la scorsa settimana a Torino si è tenuto il G7 e purtroppo nelle giornate di venerdì e sabato le manifestazioni che hanno interessato le città di Torino e Venaria sono, come era facilmente prevedibile, sfociate in violenze da parte dei soliti noti gruppi organizzati, che sono purtroppo una presenza Stefano *(PD)*. Sabato, durante il corteo che si è concluso a poche centinaia di metri dalla reggia di Venaria, il centro sociale Askatasuna, noto a tutti ed alle cronache nazionali per la sua capacità di inquinare tutte le manifestazioni pacifiche, si è reso protagonista di violenze che hanno portato all'arresto di uno dei *leader* del centro - peraltro oggi prontamente scarcerato e messo a dimora obbligatoria nel suo paese

alcuni altri capi o capetti di questo centro sociale che in queste ore, dopo aver scoperto che i giornalisti de «la Repubblica» avevano messo a disposizione il filmato sulla base del quale la polizia e la magistratura hanno provveduto all'arresto differito, come previsto dalle nostre leggi, della persona che aveva picchiato, o che avrebbe picchiato il poliziotto, uno di loro con un post su Facebook ha minacciato i giornalisti di questo quotidiano, dicendo che da questo momento verranno trattati come i poliziotti della scientifica. Conoscendo l'idea che hanno della polizia

tale Lele Rizzo - potrebbero poi produrre i propri effetti nel tempo. Mi rivolgo - ripeto - al Ministro dell'interno perché credo che la città di Torino non meriti di avere continuamente sulle cronache nazionali la propria immagine sporcata da questi centri sociali.

Tre mesi fa il sindaco, utilizzando fondi del Comune, ha fatto causa ad alcuni consiglieri comunali di minoranza, accusandoli di diffamazione nei confronti del Comune

minoranza. Stasera il sindaco chiede al Comune di votare l'incompatibilità dei consiglieri comunali di minoranza in quanto in causa con il Comune. In pratica, la maggioranza estromette la minoranza, promuovendo una causa contro la minoranza, per poi contestare l'incompatibilità di chi subisce questa anomalia. Facendo così, signor Presidente, noi faremo stare zitti tutti i consiglieri comunali di minoranza di tutt'Italia, perché basterà criticare l'operato di un sindaco affinché questo, utilizzando soldi dei cittadini di quel Comune, quindi di cittadini italiani, farà causa ai consiglieri comunali di minoranza per poi farli stare zitti, in modo da

Signor Presidente, intervengo oggi in quest'Aula per denunciare una situazione grave che coinvolge il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Sono noti i tagli che soprattutto questo Governo ha effettuato nei confronti degli enti locali e le difficoltà enormi che i Comuni hanno nell'erogare servizi ai propri cittadini in mancanza delle risorse provenienti dallo Stato centrale. Ma quello che sta accadendo in questo Comune è davvero paradossale. Dovete sapere, infatti, che il Comune di Santa Maria Capua Vetere vanta un credito di ben due milioni di euro per l'IMU (l'imposta sugli immobili), da parte di un soggetto che, nel periodo tra il 2004 e il 2009, non ha versato quanto dovuto. Allora voi mi direte: rivolgetevi ad Equitalia, fate pignorare e fatevi pagare. Purtroppo, però, il soggetto debitore in questione è la Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, nel periodo 2004-2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzò l'impianto Stir locale durante l'emergenza dei rifiuti. La Presidenza del Consiglio si è rifiutata di pagare queste somme dicendo che era un'attività svolta per fini istituzionali, per cui si è andati anche per le vie legali. Ciò fino a quando è intervenuta la sentenza definitiva della Corte di cassazione, che nel 2016 ha accolto i ricorsi del Comune di Santa Maria Capua Vetere ed ha riconosciuto l'obbligo della Presidenza del Consiglio di pagare l'imposta comunale per il periodo 2004‑2009, ed ha anche accertato che l'impianto fin dal 2011 veniva utilizzato per attività di tipo industriale, per scopo di lucro da SpA e sicuramente da soggetti diversi dallo Stato. A questo aggiungiamo, fra l'altro, che il Comune di Santa Maria Capua Vetere, dopo la sentenza della Corte di cassazione, tramite Equitalia si è attivato per la riscossione di quanto è nel suo diritto. Ma ad oggi, a distanza di un anno e mezzo, la Presidenza del Consiglio risulta ancora inadempiente. Le cartelle sono state emesse da Equitalia nel 2012 per un importo di 1.921.380 sollecitate nel 2013, ma ancora neanche un euro è stato versato. Se a questo aggiungiamo che lo stesso Comune vanta un credito da parte del Ministero della giustizia per le spese sostenute per gli uffici giudiziari nonché per il pagamento di tributi, per circa un decennio,

una legge che questo Parlamento ha varato per quanto riguarda l'IMU, ma non si attiene neanche alla sentenza della Corte di cassazione, quindi ad una sentenza definitiva. Chiedo pertanto che la Presidenza del Consiglio e il Ministero della giustizia provvedano immediatamente a pagare i propri debiti perché il Comune di Santa Maria Capua Vetere non può e non deve più sostenere questa situazione. *(Applausi

e cioè che un deputato, quindi un nostro collega in Parlamento, tale Caruso, espressione di una forza politica che si chiama Democrazia Solidale-Centro Democratico si permette di far lavorare al proprio servizio, inizialmente come stagista e poi non si sa come, una ragazza che per un anno e mezzo circa, stando a quello che è stato prodotto, risulta non retribuita. Proprio bella questa democrazia solidale nei confronti di chi lavora! Ma la cosa ancor più divertente - e mi rivolgo soprattutto alle colleghe è che questa ragazza, nella nota trasmissione «Le Iene», ha mostrato anche un messaggino che le sarebbe stato mandato, appunto, da tale deputato, in cui,

del sottosegretario Rossi.

tutte le donne italiane dovrebbero sentirsi indignate, a maggior ragione se lavoratrici, visto che il lavoro viene fatto oggetto di scambio con profferte di questa natura - sempre che sia vero quel messaggino

dei suoi dipendenti da Roma a Milano. Fermo restando che c'è una sentenza della magistratura intervenuta il 22 agosto, in cui si intima a Sky di rispettare

quantomeno inquietante il comportamento di qualche rappresentante sindacale, che forse si è dimenticato che era suo compito difendere i lavoratori e raccordarli all'azienda affinché il diritto al lavoro non venisse calpestato. Tant'è che solo alcune forze sindacali hanno levato e fatto

tale vertenza, perché è inaccettabile che, a fronte di un intervento della magistratura, qualcuno, semplicemente perché ritiene di essere grosso, se ne freghi. La legge è uguale per tutti.

Signor Presidente, la mafia è una malattia sociale che ha forma di potere, forma di potere che mira a governare le relazioni sociali; la mafia è sempre riconducibile e connessa a due elementi: terra e fuoco. Con queste parole, pronunciate dal professor Nando dalla Chiesa, è cominciata la settima edizione della Summer school organized crime 2017, con il sottotitolo: «La mafia oggi». Ebbene, in Lombardia il fuoco continua a intimidire amministratori locali e imprenditori, soprattutto quelli legati al ciclo del trattamento dei rifiuti e alle imprese edili. Ho qui un elenco di circa 25 eventi incendiari raccolti dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle nel solo anno 2017.

fare tutto quanto in suo potere affinché le procure vengano dotate dei mezzi che richiedono da numerosi mesi, se non anni. Faccio seguito anche alla richiesta della dottoressa Zanetti, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Monza, che chiede da diverso tempo almeno tre magistrati.

viene dedicato un convegno dalla Fondazione che porta il suo nome. In questa sede vorrei ricordare soltanto il sodalizio che legò Giuseppe Pera ad altri due grandi giuslavoristi

è uno sguardo molto disincantato sulla vecchia dogmatica giuridica, un po' muffosa e autoreferenziale. Questo sguardo disincantato, che ha poi segnato tutta la cultura giuslavoristica successiva, italiana e non solo, ha indotto Gino Giugni a dare valore allo studio dell'intreccio fra ordinamento statale e ordinamento intersindacale, tra fonte legislativa e fonte collettiva, tra diritto del lavoro e relazioni industriali. Federico Mancini ha valorizzato lo studio dell'intreccio tra diritto del lavoro e politiche del lavoro, poi fra diritto e politica *tout court*. Giuseppe Pera ha invece tradotto quello sguardo disincantato sulla dogmatica tradizionale in una sorta di ribaltamento del discorso giuridico. Invece di ragionare per concetti, individuando la nozione astratta e poi riconducendo ad essa la fattispecie concreta, Giuseppe Pera è sempre partito dalla ragion d'essere concreta della norma, cioè dall'interesse protettivo reale (*lato sensu* politico) da cui essa è nata, e lo ha confrontato con l'interesse in gioco nel caso singolo. A Pera non interessava un diritto del lavoro dedotto in via sillogistica dai massimi sistemi, ma soltanto un diritto del lavoro terragno, sporco di olio e di fuliggine, nel quale il buon senso del «buon giudice del lavoro» conta molto di più della logica astratta. A lui, come agli altri due giuslavoristi dei quali ho fatto cenno, deve molto non soltanto, come è ovvio, la comunità giuslavoristica, ma anche l'intero nostro Paese.